Devo solo lamentare, se il Presidente me lo consente, che la prima, quella che vede come primo firmatario il senatore Centaro e che è sottoscritta da una quindicina di senatori, reca la data del 12 ottobre 2006,

siamo occupati nell'interpellanza, siano ancora vivi, altrimenti essa non avrebbe più motivo di essere. Se però il Governo cercasse di stringere i tempi delle risposte alle interpellanze saremmo tutti più tranquilli.

sostituto procuratore a Catanzaro, e, la seconda, il procuratore aggiunto Mario Spagnolo e lo stesso De Magistris. Su questo De Magistris è stata

di 11 pagine di misfatti e di accuse precise e non mi ricordo che di questi misfatti e di tali accuse si sia mai parlato nel corso della passata legislatura;

Piuttosto che dilungarmi ora - vedremo poi nella replica - sugli elementi qui citati, vorrei ricordare al Governo che quando la relazione degli ispettori parla di «maleodorante verminaio», riferendosi agli uffici della procura di Catanzaro, questo termine - è una considerazione che sarà opportuno fare - si può tranquillamente estendere a tutta la situazione dell'amministrazione della giustizia in Calabria (e per ora fermiamoci alla Calabria). Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordo che la magistratura calabrese

Il suo portavoce in quell'occasione fu il sostituto procuratore

Quando l'avremo azzerata e gli attuali studenti delle scuole medie ne avranno preso il posto, allora potremo dire di aver fatto veramente pulizia». Devo dare atto a Pennisi e ai suoi colleghi che hanno mantenuto la parola e che in questi dodici anni hanno azzerato la classe politica calabrese.

saprà benissimo, perché prima di occupare giustamente il posto che occupa è stato un valente avvocato ed ha partecipato ad una grande quantità di processi,

Ci furono centinaia e centinaia di intercettazioni, di pedinamenti, una spesa enorme per il bilancio dello Stato e mandati di cattura. Ad un certo momento la documentazione raccolta assunse una tale proporzione che non ci fu più la possibilità di mantenerla a Palmi,

per l'assoluta assenza della minima possibile traccia di reato. Successivamente

Arrivò a Roma - l'ho anche conosciuta, mi pare che si chiamasse Omoboni - una sostituta che non era calabrese, ma era delegata per Il nostro attuale presidente Berlusconi si dovette precipitare all'alba al Quirinale, dove trovò il Presidente della Repubblica in pigiama. Il Presidente della Repubblica intervenne e le liste di Forza Italia non furono sequestrate. Durante la campagna elettorale, poi, vi fu un tentativo di incriminare due candidati di Forza Italia, Vittorio Sgarbi e Tiziana Maiolo, con l'accusa di voto di scambio. Anche questa vicenda fu fermata in tempo e non se ne parlò più.

Nell'ambito di queste operazioni furono arrestati il principe Alliata di Monreale e un'altra cinquantina di persone. Il principe Alliata di Monreale, che era avanti negli anni e piuttosto malandato di salute, fu liberato, essendo stato scagionato da tutte le accuse, in tempo per andare a morire a casa. Successivamente

gli eventuali imputati e i giornalisti. In questa operazione di Reggio Calabria fu chiuso il giornale locale, con l'accusa di essere l'organo della Massoneria,

Furono immediatamente coinvolti i politici. Dopo gli avvocati e i giornalisti, infatti, il principale bersaglio della magistratura calabrese in questi quindici anni sono stati gli uomini politici.

il coordinatore, ancora attuale, di tutte le operazioni antimafia della Calabria fu accusato di aver falsificato una sentenza. Da un'ispezione ministeriale risultò che l'accusa aveva firmato una sentenza in un paese distante 260 chilometri da Reggio Calabria, in un giorno in cui risultò in udienza a Reggio Calabria. Purtroppo, il reato, come tale, era andato in prescrizione, ma ci si sarebbe aspettati che, quantomeno, il Consiglio superiore della magistratura intervenisse sul piano disciplinare.

quando si stancano di perseguire gli avvocati, i giornalisti e i politici, i magistrati calabresi si accusano tra di loro. Vi sono procuratori della Repubblica di una città che accusano i procuratori della Repubblica di un'altra città; vi sono sostituiti procuratori che accusano per iscritto, con esposti al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il proprio procuratore, sostenendo che è un autocrate; vi sono procuratori che accusano i propri sostituti. Mi pare che si chiami Mollace un sostituto che è stato accusato dal suo procuratore, con documenti scritti, perché, oltre ad occupare abusivamente il posto nella direzione antimafia locale (oltre gli otto anni prescritti dal CSM), si rifiutava di consegnare i documenti dei processi che aveva in gestione al procuratore che glieli richiedeva e, soprattutto, continuava a gestire i cosiddetti pentiti. Il Consiglio superiore della magistratura ha finto di intervenire in tutti questi anni, sulla base delle denunce di magistrati che accusavano altri magistrati, ma non ha fatto assolutamente mai niente di serio. La cosa più clamorosa mi pare sia accaduta l'anno scorso; si sono avvicinati molto, finalmente, ad un atto di giustizia. Però - qui non è questione di destra o di sinistra metà del Consiglio superiore della magistratura voleva cacciare il procuratore di Reggio Calabria e difendeva il procuratore di Catanzaro, l'altra metà voleva cacciare il procuratore di Catanzaro e difendeva quello di Reggio Calabria.

Spero che il Sottosegretario abbia inquadrato le risposte del Governo in questo contesto, che il Ministro della giustizia non può non conoscere. In attesa della risposta, rinvio

indubbiamente la fotografia che ci ha consegnato il senatore Iannuzzi nel suo intervento corrisponde, direi per difetto, alla realtà calabrese. Regione che sappiamo benissimo essere di confine, su un crinale estremamente a rischio, con presenze malavitose ampiamente diffuse sul territorio, e che necessiterebbe, nell'interesse dei cittadini, la presenza di una magistratura attenta e non in perenne conflitto, così come almeno da tre lustri (forse anche da quattro) reiteratamente avviene. È un dato oggettivo che sin dagli inizi degli anni Novanta si cominciò a parlare di «verminai» a Reggio Calabria; poi di «verminai» si è parlato a Catanzaro. Indubbiamente queste espressioni, che evocano altre situazioni, come quelle di Messina, dove fu usata la medesima espressione, rappresentano un *vulnus* che può diventare mortale per la giustizia nel nostro Paese, e quindi nella Regione calabrese. La risposta che fornirò probabilmente deluderà il senatore Iannuzzi, perché sarà tecnica ed ancorata alla specificità delle domande.

Con le interpellanze in discussione i senatori Centaro, Iannuzzi ed altri interroganti lamentano condotte che il dottor De Magistris, sostituto procuratore della procura della Repubblica di Catanzaro, avrebbe posto in essere nell'espletamento della sua attività professionale. In linea più generale, muovono censure all'attività professionale di altri magistrati della procura di Catanzaro. Ciò premesso, si può riferire che negli accertamenti compiuti dall'Ispettorato generale e riassunti nella relazione del 12 ottobre 2005 relazione che aveva ad oggetto la posizione di magistrati diversi dalla persona del dottor De Magistris (quella ispezione riguardava più in particolare il dottor Spagnolo) - pur essendo emersi profili di irregolarità nella gestione dell'ufficio giudiziario ed aspetti di conflittualità nei rapporti interpersonali tra i magistrati stessi, il Ministro non ravvisò ipotesi tali da integrare fattispecie di illecito disciplinare e da giustificare i provvedimenti di azioni disciplinari nei confronti dei magistrati segnalati nella relazione. Si trattava di una relazione molto corposa di oltre cento pagine. Nella medesima relazione, considerate le segnalazioni, le interrogazioni parlamentari e gli esposti nel frattempo pervenuti che riguardavano il dottor De Magistris, l'Ispettorato proponeva che venisse disposta una autonoma indagine nei confronti proprio dello stesso, per poter verificare e valutare i fatti denunziati. In particolare, si faceva riferimento al contenuto dell'interrogazione scritta del senatore Bucciero, la n. 4-09170 del 25 luglio 2005, ove venivano descritte alcune irregolarità addebitabili al dottor De Magistris nella gestione di alcune indagini. In data 15 novembre 2005 il Ministro della giustizia disponeva una apposita inchiesta amministrativa. L'inchiesta non aveva ad oggetto, quindi, tutti i fatti successivamente indicati nell'interpellanza che oggi stiamo discutendo, quella del 12 ottobre 2006. Più precisamente, fra i fatti denunziati dal senatore interpellante costituiva oggetto dell'inchiesta disposta il 15 novembre 2005 soltanto il caso del fermo operato nei confronti dell'insegnante catanzarese Rosa Felicetti, nell'ambito dell'indagine cosiddetta "Balkangate". Trattasi di un fermo successivamente annullato dal GIP poiché il tipo di reato non consentiva la misura coercitiva. Diciamo che è uno degli errori da scuola elementare. Le altre vicende segnalate nell'interpellanza del senatore Centaro non costituivano oggetto dell'inchiesta amministrativa disposta il 15 novembre 2005. Per tali motivi il ministro Mastella, il 18 ottobre 2006, disponeva una estensione dell'inchiesta in corso alle vicende riportate nella suddetta interpellanza. In particolare, il 18 ottobre 2006 veniva conferito all'Ispettorato generale l'incarico di verificare: la vicenda della presunta violazione di norme di portata costituzionale che sarebbe stata rilevata dal GIP di Catanzaro in un provvedimento di archiviazione della posizione processuale di due parlamentari; la vicenda relativa all'analoga violazione dell'articolo 68 della Costituzione, che sarebbe stata denunciata dal senatore Giancarlo Pittelli; la vicenda dell'emissione di un provvedimento di fermo nei confronti di decine di soggetti già detenuti, non convalidato poiché motivato sul presupposto che il GIP tardava nell'emettere l'ordinanza di custodia cautelare richiesta. Posso riferire ai senatori interroganti che l'inchiesta amministrativa in questione si è di recente conclusa, con la presentazione della relazione ispettiva in data 8 marzo 2007. Tale relazione, come è regola, è stata trasmessa alla Direzione generale magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria per le valutazioni di competenza e per la formulazione delle conseguenti proposte al Ministro. Non appena perverrà la proposta della Direzione generale magistrati, il Ministro, esaminati gli atti e valutate le risultanze degli accertamenti, eserciterà doverosamente i poteri di sua competenza. Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ma purtroppo non sono in grado di dirmi né soddisfatto né insoddisfatto. Ora dipende: questa ulteriore relazione sull'ultima ispezione naturalmente non la conosco e non si può conoscere fino a quando non saranno

si tratta di vedere come finirà. Sono pessimista anche perché non più tardi di ieri pomeriggio, mentre cercavo le carte per venire ad illustrare queste interpellanze questa mattina, mi è capitata tra le mani questa notizia trasmessa dall'ANSA ieri alle ore da Catanzaro, nella quale si annuncia che si sarebbe svolta ieri (non so poi in che cosa sia consistita) una conferenza stampa indetta dal procuratore Mariano Lombardi e dal suo sostituto, il nostro famoso De Magistris. Praticamente, De Magistris aveva in corso un'inchiesta, ad un certo momento Lombardi gliela ha tolta, accusandolo di non averlo informato dell'emissione di un atto; De Magistris ha reagito accusando e facendolo immediatamente sapere, prima che a Lombardi, attraverso la stampa locale e all'opinione pubblica locale e nazionale, che Lombardi gli aveva tolto quest'inchiesta perché questa inchiesta avrebbe coinvolto o coinvolgerebbe il figlio di una signora che attualmente è la moglie di Lombardi. Naturalmente, non so chi dei due abbia ragione, speriamo di saperlo da quest'inchiesta, ma leggo qui: «Al suo arrivo al centro polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro dove si sta svolgendo la conferenza stampa, il sostituto De Magistris ha salutato il procuratore Lombardi e gli ha stretto la mano». Questo può anche passare per un atto di grande civiltà e di educazione, ma a me ricorda certe scene dei film americani sulla mafia, in cui due mafiosi che sono in procinto di ammazzarsi vanno a pranzare insieme e si abbracciano e si baciano. Lungi da me fino a quando non sapremo - se mai li sapremo - i risultati dell'ultima inchiesta che avete fatto.

resa che il programma annunciato 12 anni fa a nome dei suoi colleghi dal dottor Pennisi che, come ho detto, si è realizzato pienamente, ha prodotto alcune conseguenze in Calabria. Queste conseguenze sono molto semplici. La 'ndrangheta, che ancora 12, 13 anni fa era la mafia dei pezzenti, dei pastori che sequestravano di tanto in tanto qualcuno, lo nascondevano nell'Aspromonte e poi ne chiedevano il riscatto, è diventata la mafia più ricca del mondo e attualmente in Calabria fa direttamente politica e governa il territorio. Ciò lo si deve, innanzitutto, all'opera della magistratura calabrese perché quando in una Regione, soprattutto del Mezzogiorno, si distrugge un'intera classe politica, si distruggono tutti i partiti della prima Repubblica e non ce ne sono altri (perché i partiti che attualmente fanno politica in Calabria sono delle bagattelle, delle cose ridicole) è evidente che sul territorio resta solo la delinquenza.

Il procuratore, che attualmente ancora fa il *dom**inus ex machina* là*,* sostenne in quel processo che

che hanno distrutto i politici e la 'ndrangheta è diventata dieci, cento volte più forte. Queste interrogazioni, dunque, nel loro piccolo - il Governo ne tenga conto sono anche fatte per cercare di aprire gli occhi sulle conseguenze. Non è solo il discredito sulla magistratura che invade l'opinione pubblica, che non ci crede più ed ha ragione; le conseguenze si riverberano su tutto l'equilibrio democratico del Paese.

Signor Presidente, abbiamo una serie di fatti particolarmente gravi. Il primo è che da 114 giorni il dottor Mario Scaramella si trova in carcere in stato di arresto per motivi cautelari, inizialmente per il reato di calunnia, e in seguito per l'accusa - che da quanto è possibile sapere pare assolutamente grottesca - di avere organizzato un traffico d'armi. Il traffico d'armi sarebbe precisamente quello che lui con questa presunta calunnia ha consentito di sventare, consegnando alla polizia, alla magistratura e alle autorità competenti un gruppo di ucraini che è stato effettivamente colto grazie - lo sappiamo dalle carte inviate al Senato dalla procura - alle segnalazioni di Mario Scaramella.

effettuare un attentato, probabilmente ai danni del senatore Paolo Guzzanti, dello stesso Scaramella e di Andrej Ganchev, collaboratore di Scaramella. Queste persone vengono effettivamente arrestate

non succede più nulla in questo processo, non ci sono carte che attestino una qualche attività al riguardo. Improvvisamente tutto si risveglia quando, nel novembre 2006, Aleksandr Litvinenko (indicato

assassinato con quella che si può definire una microbomba sporca, cioè con del polonio che, dopo alcune settimane di penosa agonia, lo porta alla morte.

la morte di Litvinenko, il signor Aleksandr Litvinenko non viene mai ricercato dalle autorità giudiziarie per fornire ulteriori notizie, pur essendo, secondo quanto riferito da Scaramella, la fonte di quelle notizie notizie servite per arrestare persone in possesso di armamenti e, secondo la futura ricostruzione fatta dalla procura, la fonte della presunta calunnia di cui si sarebbe macchiato Mario Scaramella.

È nota a tutti la vicinanza di Mario Scaramella con Aleksandr Litvinenko, il quale viene colpito dall'attentato il giorno stesso in cui incontra Mario Scaramella; addirittura Scaramella viene indicato come uno dei possibili

Mario Scaramella viene interrogato sui fatti e collabora con le autorità britanniche, che lo ringraziano per l'ampia collaborazione ricevuta; viene ricoverato in un ospedale di Londra perché

se ne annuncia il ritorno in Italia. Il 4 dicembre il ministro della giustizia Mastella rilascia una dichiarazione nella quale «Chiedo alla magistratura di fare accertamenti seri prima che Scaramella faccia nomi». Credo sia anomalo che un Ministro della giustizia faccia una richiesta così specifica e per di più pubblica alla magistratura di fronte ad un caso così increscioso.

alla procura di Roma, che ne ha competenza, un'informativa in cui si attribuisce a Scaramella la responsabilità di calunnia ravvisabile nelle dichiarazioni di cui abbiamo detto. Con tempismo straordinario - che ci auguriamo sia sintomo di un generale risveglio della velocità dell'attività giudiziaria, ma mi pare che non lo sia

descritte sono contenute nella mia interpellanza, ma ho trovato su un giornale, il mensile «Area», un altro un altro fatto che coincide con questa grande sequenza: il 4 dicembre Mastella chiede che si accertino bene le cose prima che Scaramella faccia i nomi; il 6 dicembre il 6 dicembre c'è l'informativa della DIGOS; il 7 dicembre la richiesta e la concessione del mandato di arresto per Scaramella, ma il 5 dicembre

del colloquio di D'Alema con Putin non siano state soltanto le grandi questioni di politica internazionale, ma sia stato anche il caso Litvinenko e Scaramella. pertanto, un'ulteriore coincidenza. Questo è un aspetto della vicenda a proposito del quale già si rivelano molti fatti anomali. Scaramella poi, al suo rientro, sarà arrestato il 24 dicembre e tuttora è in carcere: 114 giorni per una presunta calunnia nei confronti di un personaggio, il signor Aleksander Talik - che è stato per anni clandestinamente immigrato in Italia,

che, guarda caso, sono avvenute nei giorni in cui Scaramella riferiva alle autorità le notizie su questo traffico di armi e su questo possibile attentato terroristico. Il Talik affermerà che le minacce erano dovute alla mancata restituzione di 300 euro, mentre il soggetto che ha subito le minacce riferiva, invece, che si trattava di ben altro argomento, senza specificare quale.

poiché era consulente della Commissione Mitrokhin - con il senatore Paolo Guzzanti, presidente della Commissione Mitrokhin. La prima conversazione di cui abbiamo notizia noi - ma forse ce ne sono state in precedenza - data 11 novembre 2005; ce ne sono decine di altre e la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di queste intercettazioni arriva il 26 gennaio 2007, cioè 14 mesi dopo. Durante questo periodo il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione è andato in eclissi, è come se non fosse esistito. esistito. Aggiungo che c'è un fatto particolarmente interessante: tra le conversazioni (questo è un documento che può essere addirittura trovato su Internet, per cui non rivelo nulla di riservato che riguardi la Giunta delle elezioni e delle

Da questa conversazione si attesterebbe, secondo la procura, la sussistenza del reato, di cui riferirò tra poco, senza che in atti emergano altre specifiche fonti di prova su tale delitto

Ministro si avvarrà degli strumenti che la Costituzione specificamente gli assegna, con l'articolo 107, e tuttavia ricordo il fatto

di 114 giorni per il reato di calunnia o se si conoscano altri casi di un reato di calunnia ravvisato quattordici che il testo in cui vi sarebbe la calunnia è stato messo a disposizione dell'autorità e senza che nuovi fatti siano emersi, tranne uno, l'assassinio di Aleksander Litvinenko. Riferendosi a quest'ultimo (cito alcuni articoli comparsi sul quotidiano "Roma",

gli ho detto che mi daranno l'informazione su chi è questa persona, su che cosa ha fatto, che porco è e da dove è uscita fuori». Il calunniato

venuto a morte violenta, anzi peggio che violenta, atroce e subdola, per vicende che tutto fa pensare - ma su questo cito gli organi di informazione internazionali, visto che quelli nazionali, con

l'arresto degli ucraini, che secondo Scaramella sono collegati a Talik, avvenuto grazie a notizie che Scaramella afferma di avere avuto da Litvinenko, e l'assassinio

l'ex presidente dell'IRI». La notizia è che, in tutto questo giro di informazioni, Aleksander Litvinenko avrebbe parlato anche della presunta vicinanza di Romano Prodi al KGB, i Servizi segreti sovietici. Questo aggiunge un aspetto inquietante che, proprio perché certamente quest'ultimo fatto non ha nulla a che fare con l'intera vicenda, né con l'assassinio di Litvinenko, né con l'anomala carcerazione

apertamente la Costituzione e, mi pare, soprattutto i diritti di un cittadino che è in carcere e di un parlamentare che è qui, in quest'Aula.

Nella materia delle intercettazioni telefoniche il Ministro della giustizia ha prestato grande attenzione al fenomeno della propalazione indebita del contenuto, tant'è che è stata assunta un'iniziativa legislativa in tal senso, volta a disciplinare la pubblicità degli atti di indagine e del contenuto delle intercettazioni telefoniche per garantire, da una parte, i diritti del cittadino e, dall'altra, l'esercizio del diritto di cronaca, nonché la tutela dei cittadini terzi rispetto alla materia dell'indagine. Nel disegno di legge recentemente approvato dalla Camera dei deputati è prevista una disciplina rigida della materia, con la segretazione delle conversazioni non utili alle indagini, che non avranno quindi mai ingresso negli atti conoscibili, venendo custodite in un apposito archivio segreto e riservato.

di natura penale in ordine alla custodia dell'archivio riservato, con un aggravamento di pena cospicua prevista dall'articolo 379-*bis* del codice penale l'inserimento dell'ipotesi colposa attribuibile al pubblico ufficiale che consenta la rivelazione di atti coperti dal segreto, quindi contemplando non soltanto l'ipotesi dolosa, come allo stato previsto dal nostro sistema, ma anche quella colposa,

il Ministro con il disegno di legge presentato ha inteso muoversi nella direzione sia di mantenere ferma l'ipotesi contravvenzionale dopo aver inserito l'ulteriore reato

nel codice della *privacy* un articolo 164-*bis,* che dà la possibilità al Garante di intervenire con atto ispettivo e quindi con sanzioni amministrative, quali la pubblicazione dell'illecito commesso dal commesso dal giornalista. Per quanto riguarda il tema delle intercettazioni a carico a carico dei parlamentari, nel disegno di legge non vi è nessuna ulteriore previsione rispetto alla legislazione vigente e, in particolare, all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che già prevede una compiuta disciplina per il caso in cui, nel corso di operazioni di intercettazione telefonica disposte nei confronti di soggetti che non siano membri del Parlamento, vengano intercettate conversazioni alle quali abbiano partecipato parlamentari. Tale disciplina risulta in linea con il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto impone al giudice per le indagini preliminari di richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, anche per l'utilizzazione di intercettazioni non disposte nei confronti di parlamentari, ma che, comunque, coinvolgono la loro persona, circostanza quest'ultima che può essere valutata solo successivamente alla realizzazione dell'intercettazione medesima. Infatti, se il giudice per le indagini preliminari ritiene necessario utilizzare le intercettazioni, «decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate». Qualora, invece, ritenga le suddette conversazioni irrilevanti «sentite le parti (...), ne decide la distruzione integrale Tanto premesso, per quanto riguarda la specifica vicenda giudiziaria, il procuratore della Repubblica di Roma ha riferito che, nell'ambito delle indagini disposte dalla procura di Napoli e trasmesse alla procura di Roma, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, furono effettuate intercettazioni di utenze in uso, tra l'altro, a Mario Scaramella. In tale ambito furono intercettate conversazioni intrattenute dallo Scaramella con il senatore Paolo Guzzanti. Al riguardo, la procura di Roma ha correttamente intrapreso la suindicata procedura, prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal GIP di Roma è attualmente all'esame della competente Commissione Commissione (dieci giorni dalla intenzione di voler utilizzare il contenuto). Lo Scaramella è tuttora detenuto a seguito di un'ordinanza di custodia in carcere del GIP di Roma per il reato di calunnia aggravata e continuata e di una ulteriore ordinanza custodiale per concorso in violazione della legge sulle armi da guerra. Nei confronti di entrambe le ordinanze sono stati esperiti i rimedi processuali previsti dalla legge. I ricorsi al tribunale del riesame di Roma sono stati entrambi rigettati. La procura di Roma ha anche comunicato che in ordine alla illegittima divulgazione di notizie riservate sta «procedendo per violazione dell'articolo 684 del codice penale». Per quanto attiene ai profili disciplinari, deve affermarsi che alla luce degli elementi acquisiti non si rilevano profili in base ai quali si possa ritenere l'operato dei magistrati procedenti tale da aver attinto in maniera indebita la sfera della rilevanza la sfera della rilevanza della tutela del parlamentare e quindi aver inciso sulla condotta corretta con violazione di regole sanzionabili disciplinarmente. Invero, le conversazioni intercettate tra lo Scaramella e il senatore Guzzanti sono state trattate secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Quanto alla sproporzione - punto sul quale si sono soffermati entrambi gli interroganti interroganti - tra il reato contestato e le misure cautelari applicate e la durata della custodia cautelare, deve affermarsi che non compete all'autorità politica entrare nel merito dei provvedimenti giurisdizionali, essendo essi riservati alla competenza dell'autorità giudiziaria. Per far valere eventuali motivi di doglianza sono apprestati rimedi endoprocessuali, che sono stati anche esperiti nel caso di specie. Allo stesso modo deve rilevarsi che la necessità di adottare provvedimenti cautelari in procedimenti per calunnia e sul protrarsi delle esigenze cautelari sono di spettanza dell'autorità giudiziaria. Certamente si può sottolineare che la scelta del legislatore è stata quella di consentire l'emissione di misure restrittive della libertà personale per questo titolo di reato. In conclusione, l'intervento del Ministro della giustizia sarebbe stato sicuramente doveroso se fossero emersi profili di abnormità, violazioni di legge o negligenze attribuibili ai magistrati, ma, in base alle conoscenze che abbiamo, allo stato non risultano in alcun caso tali negligenze, quindi non risultano presupposti per iniziative di tipo disciplinare. Posso aggiungere che i dati forniti dal DAP in ordine alle persone detenute per reati di calunnia attestano, alla data odierna, una presenza in carcere di 322 persone.

non ha ricevuto una risposta appagante. Lo dico nonostante abbia apprezzato il il Sottosegretario allorquando ci ha segnalato che il tema complesso delle intercettazioni ha formato oggetto di iniziative legislative che si sono fortunatamente concluse alla Camera dei deputati e che potrebbero contenere più appaganti ragioni delle problematiche complesse che su questo tema stanno attraversando settori sensibili dell'opinione pubblica. Ma la mia domanda, signor Sottosegretario, era completamente diversa. La mia domanda prendeva le mosse dalla spregiudicata divulgazione delle conversazioni intercettate, nelle quali apparivano anche conversazioni del senatore Guzzanti. La mia premessa riposava su ciò che impone la norma

deve essere sottoposta alle verifiche procedurali previste dalla legge n. 140 del 2003, perché divenga eventualmente legittima; prima è atto illegale, è atto che può essere distrutto. Non è un atto neutro, è un atto che per assumere legalità deve essere sottoposto a una procedura rigorosamente ipotizzata da una norma espressa, norma di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. È questa la domanda che ho formulato.

l'immediata secretazione, la custodia in luogo protetto delle telefonate dalle quali, senza ombra di dubbio, risultava che uno degli interlocutori fosse il Presidente della Commissione Mitrokhin, dunque un parlamentare della Repubblica? Non credo proprio, se è vero che ve ne è stata una spregiudicata divulgazione sulla stampa. Abbiamo ampiamente letto le conversazioni tra il Presidente e il suo consulente. Non entro nel merito dell'opportunità che il giornalista pubblicasse tali intercettazioni, anche se a volte un minimo di senso dello Stato imporrebbe un atteggiamento di maggiore cautela. Non è quello che mi interessa. Io ho chiesto, e la domanda va posta all'organo politico, se sono state effettuate tutte le ricognizioni necessarie per accertare con quali criteri siano stati sottoposti a secretazione in questa fase preliminare quegli atti, perché quegli atti erano illegittimi. Gli atti sarebbero diventati eventualmente legittimi nel momento in cui la Giunta per le autorizzazioni a procedere avesse consentito la loro utilizzazione. Altrimenti illegittimi restano e debbono essere soppressi. Questo è il dato, questo il tenore della mia richiesta. non posso escludere che in sede interpretativa l'atto illegittimo possa essere equiparato anche all'atto per il quale sia stata disposta la soppressione: se un atto è illegittimo, debbo pensare che deve essere soppresso. Bene: il regime sanzionatorio per chi pubblica atti destinati alla soppressione è severissimo. Ho posto una domanda: risulta che qualche ufficio giudiziario - e questo all'organo politico si può chiedere - abbia avviato avviato iniziative giudiziarie avverso questa situazione anomala, così clamorosamente anomala? Devo dire, signor Sottosegretario, che la sua risposta non mi ha appagato: mi dichiaro insoddisfatto anche se resto comunque

ringraziare il Sottosegretario, avvocato Li Gotti, per le informazioni che ci ha fornito. Purtroppo però non si è andati al cuore del problema. Il senatore Valentino ha sottolineato un aspetto: se c'è un responsabile, se la legge legge dà disposizione al magistrato di segretare certi documenti, qualora essi finiscano addirittura sui giornali, ci dovrebbe essere una responsabilità. Non possiamo condannare qualcuno

opportunamente citato articolo 6 della legge n. 140 del 2003 certo risponde all'articolo 68, comma

Lo stesso articolo 6 prevede che i testi delle intercettazioni e le intercettazioni stesse possono essere distrutti anche su istanza del parlamentare. Ma come fa il parlamentare a fare istanza, quando per quattordici mesi non ha saputo di essere intercettato, non ha saputo che erano in corso queste intercettazioni? Il senatore Guzzanti è stato intercettato fin dal novembre 2005 - e a quanto pare le conversazioni sono state ritenute interessanti, tant'è vero che ci si chiede di poterle utilizzare ma personalmente non è mai stato sentito, neanche dopo la fine di queste intercettazioni. Questi magistrati che giacciono per mesi nell'inattività totale non

ho motivi di ritenere che sarà liberato oggi o domani - ma non possono sentire le persone che loro stessi ritengono interessante sentire, ovvero persino il senatore Paolo Guzzanti, e non ritengono interessante sentire nemmeno Aleksandr Litvinenko. Allora, certo non emergono, come ha detto il Sottosegretario, gli estremi per un'azione disciplinare: non emergono anche perché non è stata compiuta un'ispezione e non si è approfondito nulla. nulla. Da quello che capisco, emergono gli estremi solo se dalla procura avvertono: «Guardate che stiamo violando la legge e la Costituzione: per favore fate un'azione disciplinare»! Se l'articolo 107 della Costituzione affida al Ministro questo potere, il Ministro deve esercitarlo; non può aspettare, per intraprenderla, che gli si pari davanti l'evidenza della violazione della legge da parte di qualche organo della magistratura. Deve fare qualcosa, deve assumere informazioni, quando è in ballo la Costituzione, la vita di un cittadino e, di conseguenza, la libertà di tutti i cittadini*.

Il 27 novembre 2006 il Ministro dell'interno incaricò i vertici della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del SISDE di verificare in tempi brevi l'esistenza ai propri atti di documentazione sull'eventuale utilizzazione di persone delle Forze di polizia o del SISDE in attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul *dossier* Mitrokhin o in qualche modo ad essa collegate. Il fine di tali accertamenti non era, evidentemente, di disporre alcuna attività ispettiva che potesse in qualche modo interferire con l'attività di un organo parlamentare o lederne le prerogative, bensì soltanto di poter escludere comportamenti impropri o contrari ai doveri d'ufficio da parte di appartenenti alle Forze di polizia. I rapporti trasmessi dal Capo della polizia, dal direttore del SISDE e dai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza attestano che il contributo fornito dagli organismi della sicurezza alla Commissione Mitrokhin in termini di personale è stato ridottissimo e sempre subordinato ad espressa autorizzazione. In particolare risulta che nessun dipendente della Polizia di Stato ha mai lavorato alle dipendenze della Commissione. Un ufficiale e due sottufficiali dell'Arma dei carabinieri hanno lavorato per la Commissione rispettivamente come collaboratore a tempo parziale e quali addetti all'archivio. Nel settembre 2002, a seguito di una richiesta del senatore Guzzanti, la Guardia di finanza segnalò una terna di ufficiali tra i quali individuare un collaboratore a tempo parziale non retribuito. L'ufficiale prescelto, dopo un incontro formale di presentazione con il presidente Guzzanti, non è stato mai chiamato a svolgere alcuna attività. Non vi è stato alcun rapporto tra il personale del SISDE del Servizio e la Commissione oltre a quelli intrattenuti dal direttore dell'Ufficio affari legali e parlamentari e dai suoi funzionari in occasione degli incontri con i consulenti della Commissione per l'esibizione dei documenti da questi formalmente richiesti. Il SISDE ha inoltre precisato di non aver mai avuto rapporti con Mario Scaramella e che una comunicazione in tal senso è stata resa in risposta ad una richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Inoltre, dagli accertamenti svolti non è risultato alcun comportamento di operatori delle Forze dell'ordine tendente a fuorviare o condizionare l'operato della Commissione stessa, né, d'altra parte, vi è evidenza di attività illegali di spionaggio o documentazione a danno di cittadini compiute da appartenenti alle Forze dell'ordine, in un modo o nell'altro ricollegabili alla Commissione. Si aggiunge che massima è stata la disponibilità delle Forze di polizia e del SISDE nel collaborare con i consulenti della Commissione e nel fornire gli apporti documentali richiesti, ciò che del resto era doveroso in relazione ai poteri costituzionalmente spettanti ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Per quanto riguarda i quesiti relativi all'intervista richiamata nell'interrogazione, al Ministero dell'interno non risultano elementi per asseverarne o meno la veridicità né per individuare le modalità con le quali essa è stata

come recita l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed è ben noto che i limiti all'applicazione di questo principio attengono alla sfera dei poteri dell'autorità giudiziaria e non certo dell'Esecutivo; autorità giudiziaria al cui vaglio, secondo quanto risulta, si trovano fatti e circostanze richiamati nell'interrogazione. Relativamente, infine, agli aspetti relativi alla sicurezza personale del presidente della Commissione Mitrokhin, si precisa che il senatore Guzzanti è destinatario dal febbraio 2004 di misure di protezione ravvicinata che, nel tempo, sono state rimodulate in funzione delle potenziali situazioni di rischio.

che ha avuto la pazienza e la bontà di fare le veci di rappresentante di un altro Ministero. Naturalmente ciò che il Sottosegretario ha detto ora - e di cui lo ringrazio è estremamente importante, ma se qualcuno esterno seguisse questa nostra mattinata non capirebbe nulla di ciò di cui stiamo parlando: qual era la domanda posta da me e dagli altri interroganti al Ministro dell'interno e il senso della risposta che ne è venuta. Voglio però intanto ringraziare perché è emerso un elemento positivo, importante e - direi - definitivo di cui mai prima d'ora in quest'Aula parlamentare era stata data notizia, tale che ipoteticamente possa anche essere divulgata (non lo sarà, ma comunque è un atto del Parlamento e da questo momento è pubblico). Si tratta della notizia secondo cui mai e poi mai è accaduto che funzionari di Polizia, dei Servizi segreti, dell'Arma dei carabinieri, della Finanza o di qualsiasi apparato o ufficio dello Stato, in maniera meno che legittima e scrupolosamente attestata da certificazioni - peraltro collettive, aggiungo io dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di cui mi onoro di essere stato Presidente, abbiano fatto richiesta ricevendo dall'amministrazione dello Stato l'aiuto che veniva di volta in volta domandato e che è stato espletato. In questo In questo modo il Ministero dell'interno oggi si degna di dire in pubblico ciò che finora non aveva mai detto, mentre aveva aperto un'inchiesta, che sappiamo benissimo non essere un'inchiesta sulla Commissione Mitrokhin, anzi, ricordo che il Ministro dell'interno ebbe la bontà di fare una noticina per ricordare che lui, esperto costituzionalista, non avrebbe mai commesso un errore così grossolano come quello di promuovere un'inchiesta dell'Esecutivo legislativo, su una Commissione parlamentare. Ma il punto è che la cosa fu interpretata e sintetizzata - giustamente - dalla stampa nazionale e internazionale dicendo che il Governo apriva un'inchiesta sulla Commissione Mitrokhin. Tutto ciò non ha nulla a che vedere, gentile signor Sottosegretario (che risponde anche a nome dei suoi colleghi), con la domanda che avevo fatto. la ricognizione presso i Corpi dello Stato (Polizia, Carabinieri, Servizi segreti) per vedere se essi avessero o meno illegalmente collaborato in maniera diversa da quella realizzata attraverso gli atti ufficiali e formali della legge, questa inchiesta, che è stata compiuta non sulla Commissione Mitrokhin, ma all'interno degli apparati dello Stato, fu determinata da uno e un solo articolo di giornale. dell'articolo uscito il 26 novembre sul quotidiano «la Repubblica» in cui venivano riferite parole asseritamente raccolte circa due anni prima da un certo signor Evgueni Limarev, che poi mi sono preoccupato di andare a cercare. Io, non il SISDE, non la Polizia italiana, non i magistrati, io, l'8 gennaio di quest'anno, sono andato a Cluses, armato di registratore, e ho intervistato per cinque ore questo signore, a sua volta armato di registratore. Ho pubblicato su Internet una larga parte delle cose che ha detto e ho potuto constatare che tutto ciò che aveva affermato sul quotidiano «la Repubblica» era falso, fabbricato, assolutamente inconsistente, mai detto, inventato, calunniosamente scritto contro di me. Allora la mia domanda a cui lei non ha risposto per conto del Ministro era con quali criteri il Ministro dell'interno, letto un unico e solo articolo di giornale, sulla base di questa unica notizia di un articolo, anonimo peraltro, fatto da un tizio assolutamente sconosciuto e che poi si scoprirà essere

è indifendibile quello che allora disse questo Ministro. Poi è cominciato un linciaggio a cui hanno partecipato tutti gli esponenti dei partiti, sempre sulla base di questo unico

a quanto pare - da organi dello Stato in stanze dello Stato. Questo sì è un crimine. Su questo crimine abbiamo la notizia, prima commentata dal senatore Malan come una cartellina probabilmente aperta con il caso delle intercettazioni diffuse. Credo che questo sia un evento gravissimo sul quale ancora avremo modo di riflettere, sul quale presenterò nuove interrogazioni e nuove interpellanze e sul quale il Governo sarà chiamato a rispondere. Ma sottolineo oggi il Governo non ha risposto alla domanda: con quale criterio ha fatto ciò che ha fatto e con quale criterio non ha dato pubblica notizia di ciò che ha trovato, cioè

Mi era noto che sfuggissero intercettazioni secretate. Non mi era noto però che si facessero conferenze stampa per illustrarle. Questo non lo sapevo.

l'interpellanza che oggi illustro è stata sottoscritta da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e quindi anche nella Commissione sanità e faceva seguito anche a un ordine del giorno che durante il percorso della finanziaria nello scorso mese di dicembre la Commissione sanità, nella sua unanimità, aveva rivolto al Governo affinché venisse risolta in tempi rapidi risolta in tempi rapidi la situazione degli specializzandi. Perché il problema sta così a cuore a tutte le forze parlamentari? Perché parliamo di 25.000 giovani professionisti, giovani medici

legislativo non più accettabile, in cui da un lato sono considerati come studenti, dall'altro, quando fa comodo, come lavoratori, che devono fare quindi tutta l'assistenza all'interno degli istituti clinici e degli ospedali, in una situazione oggettivamente inaccettabile e difforme dagli *standard* dell'Europa a cui pure ci siamo riferiti. Si pensi soltanto che la maggior parte di questi giovani professionisti lavora dalle 50 alle 60 ore alla settimana

Come dicevo, nel 1999 si è avviato un processo per l'adeguamento dell'*iter* formativo medico-specialistico italiano agli *standard* europei, con l'emanazione del decreto legislativo n. 368, a partire dalla normativa di recepimento di una direttiva europea sulla libera circolazione dei medici e sul reciproco riconoscimento dei loro diplomi. Da allora, purtroppo, e fino al 23 dicembre 2005 (quindi sei anni dopo), con la finanziaria del 2006, non si è fatto nulla per applicare questa legge e soltanto questa finanziaria ha introdotto il contratto di formazione specialistica che prevede che ai medici specializzandi venga applicato un vero e proprio contratto di formazione, per la cui attuazione viene indicato in quella legge uno stanziamento economico specifico e poi la posticipazione della trasformazione del loro rapporto di lavoro a partire dall'anno accademico 2006-2007. Qualcosa è successo dal momento in cui questa interpellanza è stata presentata, circa un mese e mezzo fa, perché proprio ieri la Conferenza Stato-Regioni è arrivata alla firma di un contratto, che però deve ancora passare alla fase applicativa per quanto riguarda la emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; su questo poi chiederò al Sottosegretario, eventualmente, maggiori specificazioni. Sarò sintetico, perché credo che l'argomento sia molto noto. Ci sono delle situazioni che sono emerse anche alla cronaca di questi giorni e sono state già sollevate anche in Commissione proprio dal collega Gramazio, di una circolare che è uscita al Policlinico Umberto I, in cui la direzione medica dà indicazione che vengano usati gli specializzandi in sostituzione dei medici strutturati.

non esporli a situazioni nelle quali non abbiano la piena responsabilità o possano trovarsi in difficoltà operative. A quanto mi risulta, nel contratto firmato ieri sono stati aggiunti alcuni emendamenti, uno dei quali, in particolare, potrebbe a mio avviso essere in contrasto con la norma che ho appena citato, laddove appunto si prevede che, sia pure limitatamente a a condizioni che siano coerenti con il percorso formativo, questa possibilità di sostituzione in effetti esiste. Su questo, in particolare, vista l'evoluzione della normativa, chiedo una precisazione al Sottosegretario ed eventualmente un impegno a risolvere, nei futuri passi passi istituzionali, quello che a mio parere è un conflitto legislativo che ho cercato di mettere in evidenza. La seconda parte dell'interpellanza riguarda il problema del ritardo cronico con cui ogni anno vengono emessi, da parte del Ministero, i bandi per l'iscrizione alle scuole di specialità. Pensate che in questo momento (siamo al 19 aprile) non c'è ancora il bando per l'anno accademico in corso e questo si è verificato già negli anni passati. Esistono delle normative e delle circolari ministeriali che prevedono che le Regioni (e quindi le università) dovrebbero trasmettere al Ministero il loro fabbisogno addirittura entro settembre; ciò è stato costantemente disatteso in tutti gli anni di applicazione o di pseudo-applicazione della legge. Sarebbe sufficiente che le università trasmettessero i loro fabbisogni entro la fine dell'anno, se non proprio a settembre, in maniera che i bandi possano uscire entro gennaio. Questo, come è ben noto al Sottosegretario, permetterebbe di agganciare

il Ministero dell'università e della ricerca ha avviato l'*iter* per l'applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dalla legge n. 266 del 2005. La normativa in questione prevede l'attribuzione di un trattamento economico che potrà essere assegnato ai medici specializzandi, come previsto dalla legge finanziaria 2006, mediante la stipula di contratti di formazione specialistica, a partire dall'anno accademico 2006-2007, in attuazione delle disposizioni contenute nella stessa legge finanziaria 2006, che indica uno specifico stanziamento economico. Va ricordato, in via preliminare, che la complessità dell'*iter* procedurale comporta una serie di adempimenti per la realizzazione dei quali sono necessari tempi tecnici di non breve durata. Si ricorda, infatti, che il provvedimento con il quale è stato determinato il costo dei contratti è stato predisposto da questo Ministero di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze e inviato all'approvazione del Presidente del Consiglio. Il decreto firmato è stato inviato alla *Gazzetta Ufficiale*, che provvederà alla pubblicazione dopo il controllo della Corte dei conti. Nel contempo, è stato predisposto il provvedimento con il quale è stata definita la bozza di contratto, che dopo l'approvazione del Ministero del lavoro è stata sottoposta all'esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi sarà inviato alla firma dei Ministri competenti e del Presidente del Consiglio per poi essere pubblicato. Posso comunicare con soddisfazione che la Conferenza Stato-Regioni ha concluso proprio ieri l'*iter*, raggiungendo nella prima seduta possibile l'intesa su un testo della bozza di contratto che recepisce alcune modifiche correlate, ma non identiche, a proposte delle Regioni in tema di orario di lavoro, di sostituzione del personale strutturato e di attività intramuraria. Le modifiche concordate in Conferenza per l'intesa hanno mantenuto fermo il principio che i medici specializzandi fanno parte a pieno titolo delle aziende ospedaliere universitarie, ma che ogni loro attività deve essere inquadrata nel percorso formativo universitario che stanno seguendo per il completamento della loro formazione culturale e professionale.

È da far presente, infine, che per quanto riguarda la pubblicazione del bando di concorso per l'anno accademico 2006-2007 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, la Conferenza Stato-Regioni deve esprimersi in sede di prima applicazione della nuova disciplina sull'approvazione dei fabbisogni dei medici specialistici da formare e i contingenti dei contratti proposti per ciascuna tipologia di specializzazione. Anche in questo caso la Conferenza Stato-Regioni ha dato ieri il suo assenso sui numeri totali degli specializzandi da ammettere alle scuole e sui criteri di ripartizione tra gli atenei e le relative scuole di specializzazione. È comunque impegno del Ministero quello di chiudere al più presto e positivamente sia il troppo lungo *iter* di applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, sia l'*iter* dei bandi di ammissione alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2006-2007, anche questi in inaccettabile ancorché cronico ritardo. Esprimo anche l'impegno del Ministero a seguire attivamente e da vicino la prima applicazione del citato decreto legislativo e a e a riportare gradualmente a scadenze normali rispetto ai tempi accademici i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. Infatti, è obiettivo prioritario della politica del Ministero quello di ridare fiducia ai giovani medici in formazione culturale e professionale che svolgono anche un ruolo assistenziale importante nell'attività delle aziende ospedaliere universitarie. Essi hanno il diritto di vedere il loro periodo di formazione-lavoro protetto da sicure norme contrattuali, equamente retribuito e sempre meglio inquadrato in un percorso formativo personale ben delineato e ben organizzato dalle università, anche secondo le direttive europee. Ciò contribuirà del resto - come indicato dagli stessi onorevoli interpellanti - alla migliore formazione dei nostri medici specialistici e quindi, in ultima analisi, alla salute di tutti i cittadini.

della sostituzione del personale strutturato da parte dei medici specializzandi, che la bozza di contratto su cui ieri è stata raggiunta l'intesa prevede possibile solo se in coerenza con il percorso formativo di ciascuno specializzando. È chiaro che si presenta un problema di lettura congiunta della norma contrattuale concordata e della legge. Vorrei tuttavia segnalare

di poter esercitare in prima persona atti assistenziali di cui hanno la responsabilità, con la presenza o con l'assenza del loro tutore, per poter pervenire, pervenire, alla fine della specializzazione, alla piena maturità professionale, che si raggiunge anche attraverso una graduale assunzione di responsabilità.

che si sono potute muovere soltanto dopo che il Ministero della salute ha fissato il contingente nazionale. Quest'anno esso è inferiore di oltre 2.000 posti su 7.000 a quello dell'anno precedente. Ciò ha causato un'ovvia difficoltà da parte delle Regioni a determinare il fabbisogno all'interno di una quota nazionale assai più ridotta, per motivazioni che certamente gli interpellanti conoscono, e quindi ha provocato un inaccettabile - come ho già riconosciuto

medici non avevano copertura per quanto riguarda la malattia, la maternità o i congedi. Ciò rappresenta sicuramente un importante passo avanti. Resta aperto il problema, che credo vada precisato ulteriormente, della presenza del *tutor*, dello strutturato, perché è sicuramente vero quello che dice il Sottosegretario, e cioè che il medico in formazione deve evidentemente svolgere un numero sufficiente di atti medici, qualunque che sia la sua specialità, per acquisire quella manualità così importante in tantissime branche della medicina. È ovvio che ci deve essere questa possibilità. Sappiamo benissimo che uno dei problemi delle nostre scuole è che a volte non c'è questa possibilità fisica, laddove non ci siano convenzioni con l'ospedale, e quindi una base sufficiente di pazienti su cui esercitare la professione.

Forse si possono concepire delle eccezioni nell'ultimo anno o nell'ultimo semestre di specialità; però ci vuole, per esempio, una certificazione del direttore che attesti che il medico è in grado di fare tutto.

ricerca*. Al fine di fornire una circostanziata risposta ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, il Ministero ha acquisito dal rettore dell'Università di Roma «La Sapienza» elementi conoscitivi sulla vicenda dell'immobile denominato Torre di ricerca. Sulla base di documenti in possesso dell'ateneo risulta che l'edificio venne realizzato nel corso degli anni Novanta dall'ex Genio civile, su un'area di proprietà del patrimonio indisponibile dello Stato, concessa in uso gratuito e perpetuo all'Università di Roma. Lo stabile, una volta ultimato, venne consegnato dall'ex Genio civile, in via provvisoria, al professor Balsano, quale presidente della Fondazione Andrea Cisalpino e titolare della cattedra di I clinica medica, in virtù dell'accordo di collaborazione stipulato tra l'Università «La Sapienza» e la Fondazione medesima con atto del 20 marzo 1987, della durata di anni dieci. Oggetto dell'accordo era la collaborazione sui temi di rilevante interesse scientifico e di particolare attualità, in riferimento soprattutto alle «malattie su base genetica, alle malattie allergiche e immunologiche, alle trasformazioni neoplastiche e alle risposte immunitarie», temi attinenti all'attività svolte da entrambe le strutture. Per il miglior esito della collaborazione, all'articolo 2 dell'accordo si prevedeva che le attività oggetto della convenzione venissero espletate nella Torre di ricerca dal personale di entrambe le strutture coinvolte, con la gestione della fondazione. Alla scadenza della convenzione è stato stipulato, il 24 novembre 1997, un nuovo atto, che ha dato però origine ad un complesso contenzioso tra ateneo e fondazione per l'uso della struttura. Le vicende giudiziarie sono attualmente definite dalla sentenza del Consiglio di Stato, citata nell'interrogazione, che ha annullato i provvedimenti assunti dall'università per l'assegnazione dell'immobile ai dipartimenti universitari e ha stabilito che l'università e il Policlinico non avrebbero diritto ad utilizzare la struttura a seguito della convenzione conclusa con la fondazione. La fondazione ha posto in essere ulteriori rivendicazioni promuovendo un giudizio arbitrale, che ha riconosciuto il diritto della fondazione stessa ad un risarcimento per la mancata disponibilità della Torre di ricerca per un periodo di tempo che la convenzione stipulata nel 1997 attribuiva ad essa. Il lodo arbitrale è stato impugnato dall'università presso la corte di appello di Roma, della quale si attende ora il giudizio. Allo stato attuale, pertanto, il Ministero non può esprimere un motivato parere in merito alla possibilità di adottare iniziative per una positiva soluzione dell'uso dei locali della Torre di ricerca, in quanto non è in possesso di elementi di approfondimento delle vicende giudiziarie che si sono svolte tra università e fondazione, considerato anche che le sentenze giurisdizionali sono favorevoli alla fondazione. Occorre ormai, peraltro, attendere l'esito del giudizio pendente di fronte alla corte d'appello.

ad una convenzione stipulata con il professor Balsano, che - non debbo ricordarlo - fu inquisito e condannato insieme a Poggiolini

pubblico, che fa parte di una struttura pubblica qual è l'università, bisogna compiere tutti gli atti necessari affinché quel bene possa ritornare in possesso dell'Università di Roma